ho appreso dell'emissione di una ordinanza da parte del GIP del tribunale di Milano, la dottoressa Forleo, indirizzata alla Camera e al Senato per poter avere la disponibilità delle intercettazioni di tre deputati e di tre senatori ai fini delle indagini in corso da parte della procura di Milano sulle scalate Antonveneta e Unipol. Innanzitutto vorrei dire che su queste scalate sono state pubblicate, nel corso di quest'ultimo anno e mezzo e a più riprese, numerose intercettazioni, non so se illegalmente fatte, ma sicuramente fuori dalla legge pubblicate. Sono state chieste dal Ministro

almeno in due circostanze, ha detto di aver svolto delle indagini interne per verificare come queste intercettazioni fossero pervenute a organi di stampa che le hanno successivamente pubblicate: sino a questo momento nessuno di noi ha notizia dello stato delle indagini da parte della procura. Vorrei allora che innanzitutto su questo primo punto, su questa prima questione, il Senato venisse informato dal Ministro della giustizia su come effettivamente stiano le cose, su quale sia lo stato di queste indagini della procura di Milano. Tornando però all'ordinanza della dottoressa Forleo, so bene che l'autorizzazione al Parlamento può essere al Parlamento può essere chiesta entro dieci giorni dalla decisione della camera di consiglio che ha deliberato di avanzare questa richiesta al Parlamento medesimo, in questo caso sia alla Camera che al Senato: a me risulta che a tutt'oggi

Però l'iniziativa del GIP di Milano, in sostanza, con la sua pubblicazione ha messo praticamente il Parlamento di fronte al fatto compiuto, io penso con una invasione di campo da parte del GIP rispetto al settore di operatività, di iniziativa dei in altre parole, come alcuni hanno sostenuto, si è nei fatti aperta una sorta di processo a mezzo stampa verso tre deputati e tre senatori. Non so, come dice qualcuno, se sia stata violata la Costituzione o, al contrario, come sostengono altri, se tutto ciò sia avvenuto nell'assoluta regolarità; so però che questa iniziativa si inserisce in un clima generale di antipolitica e di antiparlamentarismo. È il clima che fa dire, e scrivere a molti, a tanti, che il Parlamento in sostanza è composto di fannulloni, nullafacenti, rissaioli, quando va bene; l'impegno dei lavori parlamentari di molti di noi, che si svolge con normalità, a volte con fatica, è assolutamente ignorato: purtroppo, ci sono organi di stampa ed anche giornalisti che si esercitano in questa funzione. Ora, può darsi che qui ci siano pure dei fannulloni, dei nullafacenti, dei rissaioli o anche peggio; penso, però, che anche la più sferzante delle denunce di distorsioni, errori o manchevolezze da parte nostra nel lavoro parlamentare non solo sia doverosa, ma utile per correggere un modo di essere e di lavorare. Credo pure che il ruolo e la funzione del Parlamento, signor Presidente, siano intangibili per una ragione molto semplice: perché qui, piaccia o no, c'è l'espressione della volontà popolare. Il Parlamento non è soltanto la più alta istituzione democratica di un Paese, è lo specchio di un Paese, di ciò che il Paese è e di ciò che il Paese vuole, cioè della sua volontà e della sua sovranità. Il rispetto, quindi, non lo si deve alle persone, o soltanto ad esse, ma a ciò che rappresentano. Questo significa che i deputati e senatori siano degli intoccabili? No, assolutamente no, per fortuna no (per la verità, non per fortuna, ma per scelta dei padri costituenti). Ora, dei nostri errori è giusto che si risponda - errori di deputati o di senatori, errori gravi o meno gravi - e che si risponda di fronte alla legge. Ecco il punto: la legge. Scrivere in una ordinanza, rispetto a colleghi che non sono indagati di niente, - sarebbero: «consapevoli complici di un disegno criminoso di ampia portata in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario e finanziario nazionale» significa esulare in realtà totalmente dalle competenze del GIP; non solo, ma in sostanza si emette un giudizio e una valutazione che è già una sentenza e che pone questi parlamentari non di rispondere della propria innocenza, ma della propria colpevolezza. Ora, poiché sappiamo che è il pubblico ministero, e solo lui, che ha la competenza a formulare imputazioni, e poiché sappiamo che il GIP di Milano si è ben guardato dal rivolgere queste imputazioni, e dal rivolgersi direttamente al pubblico ministero, è evidente che ci troviamo di fronte a qualcosa che è assai grave e assai distorcente nel rapporto tra le istituzioni. Il giudice delle indagini preliminari, infatti, può procedere sulle richieste del pubblico ministero e delle parti private, ma i parlamentari di cui viene chiesta la disponibilità delle telefonate intercettate, non risultano né indagati, né sono indicati come indagabili dalla procura. Allora, tutte le esigenze probatorie che derivano da una indagine vanno, per carità, assolutamente rispettate. Penso che da questo punto di vista si debba fare chiarezza; per questo - come seconda richiesta - chiedo che anche su tale questione intervenga il Ministro della giustizia e riferisca al Senato della Repubblica, non senza però, signor Presidente, avere ricordato a noi stessi che su alcune di queste indagini in corso della procura, quelle che vengono definite «un disegno criminoso di ampia portata in una logica di manipolazione e lottizzazione del sistema bancario» - mi riferisco in particolare all'OPA lanciata da UNIPOL su BNL non esiste un solo atto, uno solo, che sia stato sindacato da alcun organo di controllo e neanche dalla procura di Roma, che aveva svolto delle indagini accurate a questo proposito:

alcuna irregolarità di legge o anche soltanto formale. Se fosse vera l'affermazione del GIP di Milano, significherebbe che nel disegno criminoso di ampia portata non sono coinvolti soltanto tre deputati e tre senatori, ma evidentemente anche questi organi che hanno omesso di esercitare la loro funzione di controllo e di vigilanza. Ai fini della trasparenza del nostro lavoro, della nostra rispettabilità e anche di quella dei colleghi che sono stati così inopinatamente, secondo me, coinvolti da questa richiesta, così motivata (perché

ma chiedo anche a questi nostri sei colleghi di fornire ai giudici di Milano la più ampia disponibilità a chiarire la loro posizione e a collaborare così alle indagini al fine di poter affermare la loro innocenza ma anche la trasparenza del lavoro parlamentare che essi sono chiamati a svolgere. *(Applausi dai

Il collega Angius è stato estremamente preciso nelle sue richieste; ha chiesto che il Governo, per voce del Ministro,

nella sede competente. Diversamente, se c'è qualche fatto nuovo rispetto ad altri temi è giusto che venga citato. Però è chiaro - lo ricordo a tutti - che questa usanza dell'apertura di seduta con sedute a schema libero è un qualcosa

Signor Presidente, convengo con le sue considerazioni di poco fa a proposito della necessità di garantire l'ordinato *iter* dei nostri lavori rispetto all'uso ricorrente di sollecitare l'attenzione da parte dell'Aula e del Governo intorno ad argomenti evidenziati nella cronaca politica. Però sono costretto a richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi sulla richiesta di una tempestiva presenza del Governo

realizzata dal Governo su temi rilevanti quali quelli riguardanti la materia del lavoro e della previdenza sociale. Si tratta - come è noto - di un documento molto impegnativo a proposito del quale in questi giorni si è detto che il Governo non intende non intende recepire modifiche di alcun tipo. L'Esecutivo sembrerebbe in partenza intenzionato ad evitare un approfondito esame parlamentare, anzi sarebbe intenzionato a non proporre immediatamente gli atti legislativi coerenti con quell'accordo, ma attenderebbe la manovra di finanza pubblica per presentarli, presentarli, nell'auspicio di mettere il Parlamento di fronte alla scelta o di un probabile voto di fiducia o comunque di un "prendere o lasciare" rispetto a disposizioni molto complesse, che toccano la vita dei cittadini. Credo sia doveroso un intervento tempestivo del Governo per descrivere questi documenti e, allo stesso tempo, per garantire il Parlamento che i tempi e i modi con cui verranno tradotti in atti normativi saranno tali da garantire il puntuale esame

lunedì scorso, sua maestà re Zahir Shah, cui il Governo ed il Parlamento avevano conferito il titolo di "padre della patria". Nella mia veste di Presidente della Commissione esteri della Camera dei deputati, dopo il 2001 ho avuto molte occasioni di incontrare, prima che rientrasse in patria, re Zahir e devo dire che fui associato anche alla Conferenza di Bonn che ha determinato - come voi sapete - la svolta in senso democratico dello Stato dell'Afghanistan. Re Zahir Shah nel 1964 aveva già emanato una Costituzione democratica in cui riconosceva gli stessi diritti agli uomini e alle donne; aveva fatto un tessuto scolastico che dava titoli e diplomi garantiti di valore; aveva cercato di portare sulla strada della socialità, cioè di lavori utili, anche l'economia di quel Paese. Ritengo, dunque, che noi siamo impegnati, attraverso il presidente Karzai, a mantenere questa eredità che re Zahir Shah aveva lasciato al suo Paese. Purtroppo dobbiamo riconoscere che il suo rientro in patria non ha portato alcuna delle conseguenze che egli probabilmente si augurava.

Presidente, esprimo qualche perplessità sulla sua decisione, anche perché sulla questione Forleo-Istituzioni c'è stato un intervento del Capo dello Stato,

la vicenda personale di un gruppo di parlamentari, ma anche una questione molto più importante rappresentata dal rapporto all'interno delle istituzioni. Peraltro, signor Presidente, non mi sembra che un intervento così deciso ci sia stato quando l'anno scorso alcuni colleghi furono

ripeto che il dibattito - che non si avvia ad aprirsi perché non lo consentirò - è assolutamente improprio, perché gli atti sono destinati alla Giunta e qualunque tipo di intervento dell'Assemblea oggi rischia di andare ad influenzare quel lavoro. Credo fosse assolutamente opportuno il rilievo del vice presidente Angius

senatori. Mi rammarico nel ricordare che il presidente Marini si era impegnato formalmente in quest'Aula a diffondere l'articolato del testo di riforma della previdenza prima dell'approvazione

della mia cortese richiesta, prese l'impegno di rivolgere al Consiglio di Presidenza la sollecitazione a diffondere questa documentazione. Il sottoscritto non ha ricevuto alcunché, né credo sia ipotizzabile informare i colleghi che i Capigruppo hanno ricevuto la documentazione nel lasso di il termine della seduta di giovedì e quella di oggi, perché ovviamente nessuno era presente a Roma, soprattutto i colleghi non residenti nel Comune o nella dunque che se è vera l'informazione, come credo sia vera, riportata su tutti gli organi di stampa, i colleghi senatori non solo non hanno mai preso visione del testo sottoposto all'approvazione del Consiglio di Presidenza, ma per quanto mi riguarda solo dopo che l'avrò letto sarò in grado di dire se è un testo difendibile di fronte al Paese o meno. Testimonio l'amarezza di un senatore della Repubblica e di molti altri, che non sono stati mai informati di qualcosa che li riguarda in maniera estremamente diretta ancorché,

della specificità delle zone di montagna. Regolarmente di tanto in tanto, ad esempio negli ultimi tre giorni, da questo Governo giungono delle proposte a dir poco preoccupanti. C'è un disegno di legge, quello sui costi della politica, che - chissà perché

mentre - chi si occupa di questi temi lo sa da anni - ci si confronta anche aspramente su altri fattori che determinano la qualificazione di una zona di montagna.

è il reiterato tentativo di sopprimere o indebolire una grande istituzione delle zone di montagna come quella delle comunità montane.

dove la montagna mantiene margini di degrado e di povertà reali, anche nella nostra opulenta società, le comunità montane esercitano ancora un ruolo indispensabile per la garanzia di determinati servizi che sembrano perfino banali tanto sono fondamentali, come la scuola, i trasporti, le poste, l'assistenza sanitaria, che piccolissimi Comuni non potrebbero garantire ai loro cittadini. Da queste considerazioni derivano tre proposte. Venga, il ministro Lanzillotta in quest'Aula a discutere di cosa sia la montagna e ad ascoltare le proposte. In secondo luogo, rivolgo a lei, signor Presidente, una richiesta: creiamo una corsia preferenziale. È stato depositato, forse per una rara volta in quest'Aula, un disegno di legge, come si dice oggi*,

La vicenda riguarda il Comune di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, dove lo scellerato sindaco ha permesso di finanziare le spese legali di otto presunti stupratori stupratori in attesa di giudizio, in attesa della giusta analisi processuale della vicenda. Il Comune stesso ha voluto interagire con un'azione scellerata. Per questo ringrazio anche la senatrice Finocchiaro, che ha saltato di netto lo steccato dell'appartenenza (il sindaco di Montalto di Castro, infatti, è stato eletto nelle liste dell'Ulivo) e ha stigmatizzato con grande coraggio e con grande forza

al Ministro dell'interno una giusta indagine sulla vicenda, che ha sicuramente colto alla sprovvista molti cittadini. Credo che una sollecitazione alla Corti dei conti sia necessaria.

Ora, non è mia intenzione entrare sulla questione delle prove o delle trattative, ma solo evidenziare e sottolineare che si tratta di una vittoria della comunità internazionale contro la pena di morte. Infatti la comunità internazionale si è mobilitata per raggiungere questo traguardo, questo obiettivo. Si è mossa l'Europa, la commissario europeo per gli affari internazionali Ferrero-Waldner, il Regno Unito, il Ministro degli esteri tedesco, la Francia, anche con la capacità di esprimere un simbolo della preoccupazione umanitaria, e il nostro Paese, con il Governo, il Parlamento nonché le organizzazioni non governative e la società civile.

una risoluzione alle Nazioni Unite per la moratoria e comunque la cancellazione della pena capitale nel mondo. Mi auguro che il Governo ci tenga informati per fare in modo che

con una sottolineatura, però, di una chiave di lettura che non riguarda soltanto la questione contingente e di merito, seppure di grande rilievo considerati i temi trattati. Il senatore Angius ha utilizzato, in relazione ad una questione altra rispetto a quella che voglio sottolineare, un riferimento alla centralità del Parlamento come luogo di espressione e di rappresentazione

Quando il senatore Sacconi giustamente pone il tema di un Governo che dialoga e conclude con le parti sociali un accordo così rilevante e quando si apprende dai giornali e dalle interviste che alcuni sindacalisti chiedono che si metta la fiducia

con riferimento al rapporto tra istituzioni e forme della rappresentanza, tra democrazia parlamentare e democrazia oligarchica, tra grandi questioni che il sistema bipolare pone e che devono diventare oggetto di una discussione nelle Aule parlamentari.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei e ai colleghi per commemorare una persona che in questi giorni ha dato la vita per salvare dei bambini italiani, in particolare due bambini che appartengono ad una famiglia del Comune di cui io sono sindaco. Voglio qui ricordare il cittadino bosniaco Dragan Cigan, di anni 31, in Italia da alcuni anni per lavorare come muratore. Lascia in Bosnia una moglie e due bambine di quattro e dieci anni. Domenica era a Cortellazzo e, pur non sapendo nuotare, si è lanciato in acqua senza pensarci due volte ed è riuscito a trarre in salvo una bambina, passandola ad un altro cittadino straniero di nazionalità marocchina, Rachid Hooumi, che ha completato il salvataggio. Poi è stato travolto dai vortici e ha perso la vita. Ritengo sia giusto esprimere il cordoglio

al genitore. Credo anche che vada solennemente riconosciuto il coraggio e la generosità di questo gesto di una persona che, probabilmente, dopo nove mesi che non vedeva i suoi figli, si è lanciato in acqua vedendo in quei bambini i suoi figli.

Infine, poiché egli ha salvato due bambini italiani, credo che la nostra comunità debba prendersi cura con umanità e fratellanza della famiglia che lascia in Bosnia.

per consentire di superare le difficoltà che ha incontrato Cigan Dragan, che da nove mesi non vedeva la famiglia per difficoltà burocratiche legate al rinnovo del permesso di soggiorno. Così pure alcuni familiari e conoscenti non possono oggi rientrare in Bosnia per in Bosnia per partecipare ai funerali, sempre per problemi legati al rinnovo dei permessi di soggiorno. Credo che il modo più giusto per onorarne la memoria sia quello, per quanto ci compete, da parte del Governo e del Parlamento, di mettere in condizione queste persone

a fare in modo che la nostra legislazione e le nostre pratiche amministrative siano all'altezza dell'eroismo e della dignità che questa persona ha dimostrato.

che ha fatto il presidente Angius poco fa. Rispetto le decisioni della Presidenza, che so ispirate a motivazioni non di carattere episodico ma di carattere più generale, generale, però mi permetto di dire che un intervento così importante e significativo, non stagionale, che riguarda la visione con la quale ci si deve rapportare sempre rispetto alla tutela

che un intervento come quello meritava la coralità delle adesioni su alcuni argomenti e commenti su altri, rispetto ai quali le adesioni sarebbero piaggerie.

terrorismo, ci sono state anche importanti inchieste riguardanti Torino ed altre moschee esistenti in Italia, viste come palestre del terrorismo. È necessario che il ministro Amato venga a riferire su tale situazione, che apre una grande ferita ancor più sulla sicurezza degli italiani. Non si tratta di rispettare la libertà di culto o di religione,

Presidente, sarò rapidissimo, ma voglio lasciare traccia del mio apprezzamento per quanto detto senatore Angius. Come ha detto l'amico Biondi, vorrei che su quel tono e su quegli argomenti vi fosse davvero un dibattito franco e serio, perché la nostra Repubblica sta vivendo un momento drammatico. L'antipolitica che si va diffondendo è figlia anche di una certa cultura che è stata diffusa e incoraggiata

dell'altra parte politica, ma è una cultura che io definisco dell'irresponsabilità, che ha reso questo Paese ormai ingovernabile. pertanto arrivato alla convinzione che non ci sono riformette capaci di risolvere i mali di questo Paese: ci vuole qualcosa di molto forte forte e molto valido. Mi fermo qui, Presidente, ma intendevo sottolineare questa parte del discorso del senatore Angius.

provvedimento sulla pressione delle gomme delle biciclette, ma il disegno di legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto, che è stata anch'esso

di mezz'ora e questo spazio di tempo venga riservato agli interventi fuori ordine del giorno; dopodiché, all'ora canonica, cascasse il mondo, si inizia a lavorare

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, credo sia sia necessaria un'introduzione di carattere più generale rispetto alla relazione puntuale che accompagna il disegno di legge, così come è stato esitato dalla Commissione affari costituzionali.

perché non sfugge a nessuno (non c'è bisogno che lo ricordi) l'importanza, la delicatezza dell'organizzazione di un sistema di informazione per la sicurezza, che non può mancare in qualsiasi comunità organizzata. L'esigenza di intervenire sui nostri Servizi segreti è sotto gli occhi di tutti, tant'è che nella passata legislatura si provò a formulare una proposta di modifica di modifica che interveniva in maniera non radicale sull'organizzazione, introducendo il sistema delle garanzie funzionali e riformando il modello del segreto di Stato. vicenda parlamentare, che nel Senato si concluse con un voto di larga maggioranza, si arenò alla Camera. Nel frattempo, i problemi connessi al sistema della sicurezza del nostro Paese non solo sono rimasti quelli

su un argomento - ripeto - così sensibile e delicato, che ha offerto sempre lo spunto per contestazioni, demonizzazioni, critiche e contrasti. Mi auguro che in

avuto ed ha qualche critica da muovere al provvedimento. Molti di noi possono avere in mente un modello diverso del sistema di sicurezza, però questo modello, qualunque esso sia, non può sfuggire a due requisiti fondamentali: deve essere un modello unitario, non solo in termini di efficienza del sistema

ha queste due caratteristiche, cioè riesce a coniugare una maggiore efficienza del sistema di informazione per la sicurezza

viene incardinata la responsabilità nella massima autorità politica di Governo che è il Presidente del Consiglio. Che significa questo? Significa che la frammentazione e la frantumazione delle responsabilità del sistema dell'*intelligence* viene a cadere.

un ulteriore organismo che è la segreteria generale del CESIS che coordina i Servizi con pochi poteri e che fa riferimento al Presidente del Consiglio.

degli uomini, dei burocrati, dei politici cercare di difendere il proprio campo di attività da quelle che si ritengono interferenze altrui. Quando due Servizi, come quelli attuali, SISMI e SISDE, fondano la ripartizione su concezioni ormai superate nel sistema dell'*intelligence* evidente che queste sovrapposizioni e queste situazioni di frizione possono non solo aumentare, ma anche paralizzare l'attività o l'efficienza dell'attività dei Servizi

la previsione che uno dei due Servizi si occupi della materia all'estero e l'altro svolga la propria attività all'interno e che il dipartimento abbia una funzione più efficace, più forte, più determinante nello stabilire anche i possibili punti di contatto che possono esistere tra i due Servizi (che devono essere punti di collaborazione e non di frizione)

anche più responsabile perché esiste un riferimento preciso, univoco nella figura del Presidente del Consiglio con tutte le garanzie che possono esserci nel caso in specie. Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che le ricette possono essere diverse, ma possa essere una ricetta assolutamente migliorativa della situazione oggi esistente. poi altre due tematiche sulle quali si cercò di intervenire anche nella passata legislatura che il disegno di legge mira a realizzare ed attuare la prima delle quali è quella delle garanzie funzionali. Le garanzie funzionali non sono altro che delle esimenti che consentono agli operatori dei Servizi di svolgere la propria attività senza incorrere continuamente nelle maglie del codice penale, che pure sono maglie chiaramente necessarie per garantire la convivenza civile, ma che possono essere assolutamente impeditive di qualsiasi attività che voglia acquisire informazioni per la sicurezza dello Stato. Le garanzie funzionali rappresentano un campo esplorato, realizzato in altri sistemi di *intelligence* e si traducono nell'autorizzazione specifica che il Presidente del Consiglio, nella sua responsabilità politica ed istituzionale, effettua nei confronti degli operatori dei Servizi che non incorreranno più nelle sanzioni penali perché quell'attività diventerà attività lecita. Naturalmente, non tutte le attività diventeranno lecite, perché vi sono una serie di esclusioni che giustamente portano i reati più gravi, che più preoccupano la società e la convivenza civile, al di fuori di questo meccanismo. Non vi potrà mai essere, per usare un termine noto alla fumettistica e alla nostra cinematografia imperante, una licenza di uccidere per un agente segreto: potrà esservi magari una licenza di acquisire informazioni con intercettazioni ambientali o di altra natura senza senza ottenere l'autorizzazione del magistrato ma ottenendo l'autorizzazione dell'autorità politica. Credo che sulle garanzie funzionali la Camera

dei Servizi segreti non tanto di un'aura di mistero romantico, ma più spesso di accuse che si possono naturalmente non condividere ma che comunque hanno albergato in tanti nostri amici della politica che oggi magari sono pronti a votare un provvedimento che finalmente metta fine a questa specie di *capitis diminutio* nella quale si dibattono i nostri Servizi segreti. Il secondo aspetto secondo noi fondamentale,

si potrà, dopo un lungo periodo di tempo e non un'eternità, accedere alla conoscenza delle vicende della nostra vita in comune nel territorio del nostro Paese. Nella Commissione, signor Presidente, si è avuta consapevolezza di questo, si è fatto un lavoro - credo - di grande responsabilità, partire dal presidente Bianco, per non parlare del correlatore, il collega Sinisi, che non so se vorrà intervenire subito dopo di me o in sede di replica, ma credo che tutti i componenti della Commissione abbiano lavorato considerando che questa riforma, così vitale per il nostro Paese, se Paese, se viene licenziata da quest'Aula con modifiche puntuali e precise, che non alterino il disegno complessivo e che non siano anche numericamente eccessive, potrà avere forse un via libero definitivo dalla Camera con una ulteriore lettura; se così non fosse, ritorneremmo al ping pong parlamentare e forse questa riforma, che comunque noi riteniamo utile per il Paese, potrebbe vedere la luce troppo tardi, oppure non vederla mai. Per questo anche la linea dei relatori, confortata dalla dalla linea assunta in Commissione dalle forze politiche presenti, è una linea di prudenza nella modifica del testo, anche se non vi potrà sfuggire

generale.Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, era ed è, certamente e finalmente, giunto il momento di porre mano ad una nuova riforma della legge n. 801 del 1977, in materia di organizzazione dei nostri Servizi di sicurezza e di regolamentazione del segreto di Stato. Di fronte ai ricorrenti e alle volte gravi o addirittura gravissimi scandali ed episodi criminosi che hanno coinvolto, anche dal 1977 in poi, appartenenti ai Servizi segreti italiani, si è spesso parlato di Servizi segreti deviati. Una delle ultime volte in cui ciò è successo risale alla settimana scorsa, quando, in relazione alle nuove indagini sulla strage di via D'Amelio a Palermo del 1992, è stata nuovamente utilizzata l'espressione «Servizi segreti deviati». Ma questa è una formula che lascia il tempo che trova e che non rappresenta assolutamente la realtà dei fatti. Lo diceva lo stesso procuratore nazionale antimafia alcuni giorni fa, a proposito appunto della strage di via D'Amelio. Lo andiamo ripetendo purtroppo da molti, da troppi anni. Proprio perché la ripetitività di certi episodi e le analogie con comportamenti per così dire vecchi e datati, qualcuno addirittura di vari decenni fa, congiuntamente alla carenza di verità e di trasparenza, hanno ingenerato sempre maggiori perplessità e sospetti. Tanto da far dubitare che si possa davvero parlare di "deviazione", sembrando piuttosto che alle volte ci si trovi innanzi al comportamento ordinario dei Servizi segreti, che quando rispettano norme e disposizioni e quando collaborano con polizia e magistratura allora sì paiono deviare dalle loro ordinarie procedure comportamentali. Pur affermando questo, non può certamente essere dimenticato però che, negli anni, ci sono state operazioni anche brillanti poste in essere dai nostri Servizi di sicurezza. Come non va dimenticato che sarebbe quanto meno ingeneroso, se non proprio errato, dare un giudizio negativo, assoluto e generale, su di loro e in special modo su tutti i singoli appartenenti al SISMI o al SISDE. Zone d'ombra, e peggio, ci sono state (la scoperta recente del covo di via Nazionale di Pio Pompa ne è la dimostrazione). Ma ci sono state anche vicende positive e rassicuranti (come quelle relative al reparto addetto alle missioni all'estero). Ciò non di meno, se giacciono in Parlamento da molti anni diversificati progetti di legge di modifica e di riforma, significa che da più parti si è avvertita e si avverte la necessità, sempre più pressante, di dare una risposta nuova, in termini di chiarezza e di legalità, con particolare riferimento alla esigenza di impedire (o almeno di limitare) abusi e sorprusi in violazione della legge penale e all'esigenza di garantire una gestione del segreto di Stato più consona ad uno Stato libero, indipendente e democratico; segreto di Stato che non sia più di ostacolo all'accertamento di gravi e gravissimi fatti criminosi (come le stragi o i sequestri di persona). Per anni, fino a questa legislatura, nessuna forza politica e nessuna maggioranza parlamentare hanno avuto la forza, la capacità o il coraggio di procedere sulla strada di una riforma in materia. Non sono forse questi né il momento né la sede per approfondirne nel dettaglio aspetti e cause. Fatto sta che finalmente pare giunto il momento di procedere concretamente sulla via di una riforma. Decidendo di riformare la struttura dei nostri apparati di sicurezza, potevano essere percorse strade diversificate. E l'abbondanza di suggerimenti che provengono dai vari disegni di legge presentati sta lì a confermarlo. Un analogo discorso può essere fatto in ordine alla regolamentazione del segreto di Stato e in ordine al controllo di competenza di un organismo parlamentare sull'organizzazione e sulla gestione delle attività di *intelligence*. Il Governo e il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che ci troviamo ora ad esaminare, si muovono, a mio parere, lungo una linea di sostanziale continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 in tema di organizzazione dei nostri apparati di *intelligence* e di sicurezza, anche se va dato atto di una maggiore cura e di una maggiore attenzione nel regolamentare l'istituzione, le finalità e i compiti delle nuove strutture, come va dato atto di un'impostazione istituzionale che vede affermato, in modo importante, positivo e coerente, il ruolo preminente del Presidente del Consiglio dei ministri.

ma in misura a mio parere ancora non soddisfacente) e il segreto di Stato. Ed è in particolar modo quest'ultima parte sull'opposizione del segreto di Stato quella che viene maggiormente incontro alle pressanti richieste di riforma e di verità, formulate ad ogni livello sociale e istituzionale, a partire da anni ormai lontani, quelli della strage di piazza Fontana, della strage di Bologna e della strage di Ustica. La segnalata continuità rispetto alle scelte del legislatore del 1977 si ricava sostanzialmente dalla opzione, chiara e netta, per un sistema binario, o duale, con la previsione di un coordinamento superiore:

di efficienza, di affidabilità (soprattutto democratica) e di pieno coordinamento, soprattutto rispetto ai dubbi derivanti dalla necessità di evitare contrapposizioni e sovrapposizioni (per di più, in presenza di assegnazioni di fondi sicuramente rilevanti). Contrapposizioni e sovrapposizioni, che fanno particolare riferimento sia ai rapporti (non pienamente regolamentati) con gli organismi info-investigativi delle varie Forze di polizia con competenze in materia di eversione, terrorismo e criminalità organizzata), sia soprattutto agli altri apparati di *intelligence* militare (SIOS Marina-SIOS Esercito-SIOS Aeronautica e organismi collegati), dei quali il disegno di legge al nostro esame non si occupa (a mio parere inopinatamente). In assoluto distacco rispetto al passato, la proposta di legge n. 1335 introduce *ex* *novo* una struttura molto speciale, una novità che mi pare assoluta (almeno dal punto di vista legislativo): un ufficio ispettivo, con competenze molto ampie e pregnanti e con una autonomia e indipendenza di giudizio che lo stesso testo di legge definisce "piena". Trattasi di un organismo *ictu* *oculi* molto delicato, di una sorta di servizio di sicurezza all'interno dei servizi di sicurezza. Proprio le sue peculiarità, peraltro, come argomentato anche in sede di redazione e di approvazione del parere della Commissione giustizia, necessitano di molte cautele, anche normative, in ordine soprattutto ai criteri di scelta e di formazione dei nuovi "ispettori", È ben vero che si fa rinvio ad un regolamento successivo. Ma di questo regolamento riteniamo che il Parlamento dovrebbe essere adeguatamente, dettagliatamente e preventivamente informato, senza ricorrere sul punto a regimi di particolare riservatezza, regimi sempre sospetti, in considerazione della delicatezza della questione e dei ben noti guai del passato anche recente o recentissimo. Alcuni altri aspetti del nuovo disegno di legge meritano invece ampio e convinto sostegno: *1)* quello che finalmente pone un limite, chiaro e netto, sostanziale e temporale, al segreto di Stato; *2)* quello che regola in maniera convincente l'opposizione del segreto di Stato quello sui poteri del CO.PA.CO., anche se pure a questo proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti per l'ampliamento di tali poteri, sul modello di quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta, *4)* quello che tratta delle cosiddette "garanzie funzionali" per gli uomini dei servizi segreti, garanzie contemperate da alcune disposizioni a tutela delle persone.

o lasciato in sospeso dal disegno di legge, e però foriero di contrasti e polemiche ad ogni livello istituzionale, è quello relativo alla permanenza dell'obbligo del segreto di Stato anche per una persona indiziata di reato o addirittura imputata.

siano idonee a garantire una gestione maggiormente lineare e democratica dei nostri apparati di sicurezza e siano più rispondenti alle esigenze di trasparenza, di legalità e di separazione dei poteri, così come delineati nella nostra Carta costituzionale.

Grazie, signor Presidente,

grazie per aver detto che potrebbero esservi ricette migliori,

vi è un modello unitario che individua chiaramente le responsabilità e allora vorrei che in sede di replica mi dicessero in quali termini sono definite esattamente le responsabilità di un Sottosegretario o Ministro del quale, tra l'altro, è detto che la nomina può essere eventuale o meno. Allora è chiaro che quando in un disegno di legge si prevede la possibilità di avere o meno la nomina di un Sottosegretario, che in fondo è il numero uno, in tutto il discorso, dopo il Presidente del Consiglio, si lascia tutto a mezz'acqua. Se il Sottosegretario è nominato, non è stabilito chiaramente quali sono le sue responsabilità e se non è nominato allora è inutile dire che ci può essere un nuovo Sottosegretario e le responsabilità politiche (che indubbiamente devono essere nelle mani del Sottosegretario, perché obiettivamente il Presidente del Consiglio non può gestire il discorso) non si sa bene dove andranno a finire. Aggiungo che attualmente non vi è nessuna diarchia, perché in realtà la legge vigente prevede che il luogo dei punti sia il comitato di

non è successo nella realtà; al di là delle chiacchiere e delle affermazioni di alcune persone che si autonominano responsabili e conoscitori dell'argomento, dopo tutte le accuse di deviazione non se ne è scoperta una per cui francamente abbiamo una magistratura e una polizia giudiziaria assolutamente incapaci in cinquant'anni di scoprire quanto ripetutamente denunciato, oppure possiamo pensare che le denunce fossero delle panzane. Detto questo, vi è la necessità di una nuova legge, aggiornata, per carità.

una maggiore pericolosità dovuta al più intensificato traffico di droga e di sostanze stupefacenti; vi è il fenomeno dell'immigrazione, che nel 1977 non era così violento; vi è un allargamento della criminalità internazionale; vi è la criminalità economica, che nel 1977 non era così minacciosa; vi è la criminalità ambientale relativa ad inquinamenti atmosferici, a discariche, a scorie, che allora non c'era; vi è il rischio delle attività terroristiche interne,

controllato e limitato perché vi erano i due blocchi ed il tipo di difesa era chiaramente individuabile. Di meno, per fortuna (sempre esprimendoci con cautela), vi è il rischio del terrorismo interno. Allora, nel 1977, era assolutamente prevalente questo rischio; oggi, per fortuna, seppure dobbiamo ancora piangere vittime di questa terribile minaccia, in realtà bisogna complessivamente riconoscere che essa è diminuita. Per quanto riguarda le minacce esterne, il discorso è uguale. Vi è più terrorismo; vi è la minaccia della proliferazione delle testate di distruzione di massa e dei vettori che le possono portare; vi è la criminalità internazionale, che è diventata di grande peso; vi è l'immigrazione selvaggia e l'organizzazione esterna di tale immigrazione selvaggia; vi è il rischio dell'inquinamento dell'ambiente, sia marino che aereo; vi è la criminalità economica, che rappresenta un'altra minaccia alla nostra tranquillità economica internazionale.

A ciò si aggiunge anche la necessità del controllo parlamentare che è stato ricordato e che certamente è auspicabile;

quasi dimenticato, perché sulla sua azione si deve sempre stendere un velo di riservatezza. Nella legge

Vi è la chiarezza della dipendenza e dell'appartenenza. Come è già stato accennato, le due strutture SISMI e SISDE da una parte dipendevano dalla Presidenza del Consiglio e dall'altra dai due Ministeri;

Vi erano la necessità di un controllo finanziario più puntuale, l'organizzazione strutturale da rimettere a punto, precisazioni da fare sull'arruolamento e sulla formazione e conflitti di competenza tra le varie istituzioni: queste obiettivamente erano le ragioni per le quali da quindici anni era necessario un aggiornamento della legge vigente. Molte cose sono

Vi è un migliore controllo finanziario che ritengo opportuno; sono chiariti bene i conflitti di competenza e la possibilità di adire la Corte costituzionale (rimane solo un dubbio che spero poi in discussione generale potrà essere chiarito);

Come accennato prima, si parla di un'autorità incaricata, di un Sottosegretario. Prima di tutto si dice, come già diceva la legge vigente, che la responsabilità e l'individuazione della definizione di linee di politica dell'informazione fanno capo al Presidente del Consiglio, però obiettivamente non si può pensare che il Presidente del Consiglio

spiegherò poi, che si attribuisce al capo del Dipartimento, che è un funzionario civile, la responsabilità di tutto.

In realtà si è creata una struttura binaria che però è legata mani e piedi dalla dipendenza del funzionario capo del Dipartimento. Allora abbiamo creato una soluzione unitaria, che a me può stare anche bene, Ciò che non mi va bene è che non si capisca che non si deve affidare ad un funzionario l'unitarietà, ma essa si deve affidare all'autorità politica. Invece qui il Sottosegretario rimane a mezz'acqua: quando si definiscono le responsabilità del Dipartimento e quando si parla di competenze, il Sottosegretario a volte compare e a volte non compare. Si dice invece chiaramente che i capi dei due Servizi devono riferire al Presidente del Consiglio tramite il capo del Dipartimento,

questa confusione di responsabilità e questa complicazione degli affari semplici, di trasmissione, specie con riguardo

piuttosto un'autorità politica attentissima a cui si possa accedere immediatamente, in luogo del meccanismo che è stato delineato. Desidero leggervi un passaggio per dare l'idea di quanto sto dicendo. Ad un certo punto, nel definire le competenze dell'Agenzia per l'informazione e la sicurezza esterna, e lo stesso per la sicurezza interna, si dice che «L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri». Bene, se risponde al Presidente del Consiglio dei ministri deve avere il contatto diretto con il Presidente del Consiglio dei ministri. Si dice ancora: «L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno, per i profili di rispettiva competenza».

non compromettente, non ritardante immaginare che certamente il Presidente del Consiglio (ma questo vale per tutte le norme) sia il responsabile primo; che un Sottosegretario con delega sia responsabile della gestione politica, sia capo Dipartimento e coordini, conduca l'azione di sintesi, elabori e controlli l'autorità politica e amministrativa; che il Dipartimento sia costituito da uno *staff* o da una unità centrale del Sottosegretario e poi dai due Servizi AISE e AISI, come in fondo è oggi il CESIS; che vi sia un comitato di coordinamento, in cui il Sottosegretario parla con queste tre entità (l'unità centrale di sintesi, il direttore dell'AISE e quello dell'AISI) e mette a punto tutte le azioni di coordinamento, non lasciandole ad un funzionario;

per essere stata, malgrado quanto stabilito dal Regolamento del Senato, esclusa da una competenza diretta in sede di discussione. discussione. È stato deciso così e si è assicurato che si sarebbe tenuto conto del parere importante della Commissione difesa. La Commissione difesa ha espresso un suo parere: non è stata presa in considerazione nemmeno una parola di quel parere. È un'autentica porcheria, perché non si può fare un'affermazione e poi, invece, ignorare assolutamente quello che, legittimamente e in base al Regolamento, i componenti della Commissione difesa avrebbero potuto esprimere in sede di Commissioni congiunte. Non credo vi sia una dignità di primo grado e una dignità di secondo grado tra i componenti delle diverse Commissioni. Non credo sia giusto affermare

Vorrei aggiungere che queste proposte erano oggetto non di una rivoluzione, ma soltanto di una migliore definizione di competenze, dipendenze, capacità di coordinamento e di controllo.

Per il resto confido nell'Aula e spero di essere stato chiaro: nessuna rivoluzione, ma solo adattamenti funzionali

*(Ulivo)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi in quest'Aula si discute il disegno di legge n. 1335, provvedimento che innova e riforma la normativa relativa ai Servizi di informazione per la sicurezza dello Stato, ormai superata dai mutati scenari nazionali ed internazionali e dal correlato ampio ventaglio di minacce alla sicurezza del Paese.

storico in cui riemergono logiche, da un punto di vista culturale e persino emotivo, in cui la parola "*intelligence*" viene associata a qualcosa di estremamente ostile. Oggi, come nel passato, i Servizi segreti, come percepito nell'immaginario collettivo, sono qualcosa di negativo o, peggio ancora, uno strumento attraverso il quale una parte del potere tiene sotto controllo l'altra. Ritengo che le "deviazioni", le "patologie" siano e debbano essere chiarite nelle sedi istituzionali competenti. Per contro, credo che il lavoro dell'*intelligence* debba essere al servizio e non contro il bene comune, bene comune, come strumento di difesa della Repubblica e della democrazia da qualsiasi tipo di minaccia, interna o esterna che sia, proprio nella consapevolezza che la sicurezza è un diritto di ogni libero cittadino. solo alla sicurezza su una metropolitana o su un aereo, senza correre il rischio di essere dilaniati da una bomba, ma anche alla stabilità del nostro sistema economico, alla sovranità della Repubblica e a tutto ciò che garantisce le nostre libertà. Ovviamente sappiamo tutti che l'*intelligence* rappresenta una parte del lavoro dei Servizi di informazione e sicurezza, che coincide sostanzialmente con la conoscenza, la ricerca, le capacità di analisi e di previsione. Sappiamo altresì che nell'interesse supremo della Nazione, talvolta è necessario andare non contro la legge quanto oltre la legge. Questo tema, molto serio, nel provvedimento è stato affrontato con l'introduzione dell'articolo sulle garanzie funzionali. Se, come ho detto, nel mondo dell'*intelligence* è talora necessario andare oltre la legge, è altrettanto vero che ciò non deve mai tradursi in un approccio secondo il quale tutto è sempre giustificato dal fine superiore. Quindi, l'ottenimento del risultato non deve mai essere subordinato a regole, procedure o garanzie. Dobbiamo confrontarci con quella che potrei definire la "cultura del limite", a dire che non solo ogni azione deve essere commisurata alla minaccia, ma anche che oltre alcuni limiti non si potrà e non si dovrà mai andare. Credo, insomma, che *intelligence* e rispetto dei diritti umani non siano contrapposti; al contrario, la capacità di utilizzare uno strumento così delicato nel rispetto dell'umanità, della dignità delle persone, siano pure assassini, nel medio e lungo periodo, non potrà far altro che rafforzare la capacità dei Servizi di potersi rapportare al mondo esterno. Vale la pena riflettere anche su quanto la negazione dei diritti, alla fine, non rappresenti l'origine di una minaccia ben superiore a quella che volevamo combattere. In altre parole, se Abu Ghraib e Guantanamo servono a proteggerci dal terrorismo o se non abbiano rafforzato e legittimato coloro che il terrorismo predicano e praticano. Questa è una vera sfida per l'*intelligence* del futuro. Nello stesso tempo un'altra sfida è quella di prevenire i rischi e non di trovare le giuste informazioni utili, poi, a reprimere. Prevenire, quindi, significa lavorare quotidianamente dietro le quinte senza cavalcare l'onda dell'emergenza e sviluppare anche una capacità di analisi estremamente penetrante. Tale obiettivo può essere raggiunto se questo mondo si aprirà sempre di più a quello dei saperi ed in particolare al mondo dell'università, ed in tal senso va la previsione di nuove procedure di reclutamento del personale, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, previste all'articolo 21, su cui mi soffermerò nel momento in cui si esamineranno gli articoli. Solo attraverso questo percorso, sicuramente non facile e ancora largamente da costruire nel nostro Paese, si potrà fare un salto qualitativo per cercare di comprendere in anticipo quali siano i rimedi affinché le minacce non si concretizzino. L'ultimo punto riguarda ciò che possiamo definire una "nuova cultura dell*'intelligence*", proprio perché si diffonda nell'opinione pubblica la percezione della sicurezza come tutela e non come un nemico, un golpista o qualcosa o qualcuno di cui diffidare. Condividendo quindi l'impianto ed i princìpi della riforma, ritengo siano state apportate importanti modifiche anche nel lavoro svolto nel Comitato ristretto e nella Commissione affari costituzionali al fine di migliorarne ancora l'impostazione, sotto l'aspetto di una maggiore trasparenza delle procedure, soprattutto relativamente all'esigenza di una puntuale specificazione delle disposizioni relative al personale.

Signor Presidente, colleghi senatori, molte argomentazioni andrebbero svolte su questo provvedimento di rilievo critico, per scelta, nell'interesse della chiarezza e della trasparenza. Argomenterò solo su alcuni aspetti che riguardano le linee-guida della riforma. Certamente, la materia è estremamente delicata e, giacché il rafforzamento dell'efficacia dell'*intelligence* è essenziale per la difesa in uno Stato che intende guardarsi da attacchi, sia esterni che interni. Le vicende recentissime, che hanno coinvolto settori nodali del sistema di sicurezza statale, ancora oggetto di indagine, hanno condotto in Parlamento a questo disegno di legge con una urgenza particolare; anzi, a tale proposito, auspico l'opportunità di vagliare immediatamente, a ridosso della presente riforma, il progetto di cui mi pregio di essere promotore, che intende istituire Commissioni parlamentari di controllo e di inchiesta sui *dossier* illegali SISMI, prodotti dal 2001 dal 2001 al 2006, al fine di evitare alterazioni ed inquinamenti in settori chiave dello Stato e dare continuità e prosecuzione al progetto di riorganizzazione della materia. Fondate le ragioni della necessità di addivenire alla modifica della disciplina sulla sicurezza statale attraverso un esame che sia rapido, ma approfondito ed esteso alle numerose proposte inserite nell'Atto Senato in votazione, ma sempre articolato ed esteso, questo progetto altrettanto enorme è la nostra responsabilità di cercare di superare le dispersioni di potere e gli errori del passato che non lasciano spazio ad interventi limitati e settoriali. In altre parole, dobbiamo apprezzare questa riforma, che appare omnicomprensiva e compiuta, caratteristiche tali da consentire una buona riuscita nonché un'approvazione rapida e di larga intesa. Nel dettaglio trovo pertinente l'assunto dell'articolo 1, che unifica responsabilità del sistema in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, individuato come la più elevata Autorità nazionale per la sicurezza, concessione generale della politica informativa e compiti di alta direzione. Una concentrazione di ruoli, prima troppo frazionati, che determina funzioni e compiti in maniera da costruire e definire un sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica razionale ed efficiente. Anche l'articolo 3, che introduce la figura dell'«Autorità delegata», e l'articolo 4, che istituisce il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, marciano nell'unico senso di dare alla sicurezza un sistema coeso e organico, che diventi espressione di una linea politica unitaria come unica è la finalità di salvaguardare la difesa dello Stato. Assoluta novità sono anche le disposizioni, di cui agli articoli 6 e 7 del presente disegno, laddove si istituiscono due Servizi di informazione: uno di sicurezza esterna (AISE) e l'altro di sicurezza interna (AISI), a cui vengono affidate separatamente la funzione di raccogliere tutte le informazioni utili alla indipendenza, integrità e sicurezza della Repubblica, in attuazione anche ad accordi internazionali. statuizione che è garanzia di trasparenza ed affidabilità e che riguarda la netta divisione tra i due organismi e l'ampliamento dei compiti di questi rispetto a tutte le altre articolazioni pubbliche. Da ultimo doveroso è un accenno agli articoli relativi alle garanzie funzionali, dal 17 al 20, che introducono una disciplina speciale, organica ed unitaria in tema di tutela penale del personale di sicurezza. In concreto, una disciplina che se, da un lato, ha portata integrativa nel colmare lacune preesistenti, dall'altro, si pone come accrescitiva delle garanzie per tutto il personale dell'*intelligence* statale. Si tratta cioè di scriminare penalmente alcune condotte del personale della sicurezza, talvolta lesive della normativa, purché esse perseguano finalità istituzionali. Tuttavia, condivido l'ammonimento della Commissione giustizia a vagliare bene la rispondenza ai dettami costituzionali delle riconosciute scriminanti rispetto ai luoghi e agli ambiti di applicazione delle stesse, in modo da non creare privilegi senza limiti o categorie speciali di personale. Il capitolo finale dedicato al segreto di Stato racchiude novità al passo con un sistema più moderno, coerente e adeguato alle più accreditate strutture internazionali. In buona sostanza, stimo la modifica al nostro vaglio di alto contenuto e dettata a tutela di un principio equilibrato di segreto di Stato, nell'interesse della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione.

*(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'atmosfera politica che caratterizzava l'Italia nel 1977, ricca di episodi di violenza degli opposti estremismi, non impedirono alle forze politiche, in un Parlamento caratterizzato da una forte contrapposizione ideologica, l'approvazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che definì la normativa dei Servizi di informazione e sicurezza in linea con i princìpi democratici ed i valori costituzionali. Fu una legge frutto di una straordinaria capacità di dialogo e di un'elevata sensibilità istituzionale, che permise di porre dei punti fermi a questa disciplina, al fine di poter contrastare i vari episodi di terrorismo interno che hanno caratterizzato quegli anni, che ricordiamo come gli anni più duri e più bui della nostra storia contemporanea. Nonostante tutto l'impegno e gli sforzi del legislatore dell'epoca, ben presto questa legge divenne non più adatta a fronteggiare il cambiamento politico e sociale che si venne a delineare negli anni successivi, specie dopo diversi episodi di politica estera, primo fra tutti la caduta del Muro di Berlino nel 1989. Si delineò l'idea che occorreva riformare la normativa dei Servizi di informazione e di sicurezza, ma tutto ciò non avvenne; neanche nel 2001 con l'attentato alle Torri gemelle si riuscì a smuovere le coscienze delle forze politiche. Nonostante tutti questi cambiamenti in ambito internazionale, non solo dal punto di vista geopolitico, ma anche dal punto di vista economico e tecnologico, la nostra *intelligence* ha dimostrato una buona capacità di reazione, conseguendo brillanti risultati in contesti ritenuti impenetrabili da parte di qualsiasi altro Servizio occidentale. E' arrivato il momento però di dare a questo Paese una nuova *intelligence* che stia al passo con i tempi, che sia coerente con gli scenari di sicurezza interna ed internazionale, attraverso regole più moderne, anch'esse al passo con i tempi. Tutto ciò soprattutto per permettere di fronteggiare al meglio le diverse ed innumerevoli situazioni che oggi, nell'ambito delle diverse operazioni militari, come riferito dal capo di Stato maggiore della difesa, l'ammiraglio Di Paola, in corso di audizione, sono ben diverse dalle situazioni e dalle esigenze che si riscontravano anni fa. Difatti, i rischi che oggi siamo costretti a fronteggiare sono rappresentati da possibili oppositori militari, dalla minaccia terroristica, dalle forme di impiego di armi innovative cosiddette asimmetriche o dall'utilizzo di armi di distruzioni di massa; né va trascurata la minaccia che può derivare dalla criminalità organizzata sia nazionale che internazionale. A distanza di trent'anni, solo oggi siamo riusciti, dopo un lungo e delicato confronto, a trovare il giusto equilibrio per dare una nuova e più trasparente disciplina alla materia in questione, cercando di colmare quei vuoti che negli anni hanno penalizzato la nostra attività di informazione e sicurezza. I colleghi della Camera dei deputati sono riusciti a dialogare e a confrontarsi su un argomento così delicato, distaccandosi dallo scenario politico e dai continui distinguo, ottenendo un testo normativo, frutto di una collaborazione reciproca e leale, che soddisfa le diverse esigenze di entrambi gli schieramenti politici. Anche nella Commissione affari costituzionali del Senato, sulla base del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, si è riusciti ad apportare modifiche minime ed indispensabili senza stravolgere il provvedimento in questione, al fine di mantenere il giusto equilibrio tra maggioranza ed opposizione che ha permesso di ottenere un disegno di legge che giudichiamo soddisfacente. Uno dei vuoti normativi che con il nuovo testo si andrebbe a colmare, qualora fosse approvato da quest'Aula, riguarda i rapporti tra *intelligence* e autorità giudiziaria. Infatti, gli agenti preposti alla difesa e alla sicurezza nazionale possono trovarsi a dover fronteggiare operazioni non convenzionali, ovvero possono esser costretti a dover tenere condotte tali che, normalmente, sono riconducibili alle sfere dei reati, ma che per la difesa del nostro Paese e per il perseguimento delle finalità istituzionali sono necessarie. Esempio di ciò si verifica ogni volta che un agente si introduca in modo illegittimo per impedire un possibile attentato, o che operi sotto una falsa identità, rischiando una condanna penale alla quale si può sottrarre solo ricorrendo al segreto di Stato. Con questa riforma finalmente si fa chiarezza su questo nodo normativo, dando le giuste garanzie (cosiddette garanzie funzionali) a chi, per la difesa e la sicurezza nazionale, spesso si trova in situazioni delicate e pericolose. L'articolo 17 del disegno di legge introduce, dunque, una specie di causa di giustificazione del personale dei Servizi impegnato in attività di *intelligence*, facendo comunque salvo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale. L'unica osservazione che si potrebbe muovere a tale norma, come giustamente ci è stato fatto notare in sede di audizione dall'allora comandante generale della Guardia di finanza, il generale Roberto Speciale, è che essa prevede unicamente una tutela dal punto di vista penale, tralasciando l'eventuale responsabilità in altri ambiti dell'ordinamento giuridico (civile, amministrativo-contabile, disciplinare). Sarebbe stato più equo, secondo noi, prevedere da parte nostra anche una maggior garanzia e una più ampia tutela per questi ulteriori settori. Una forma di tutela ulteriore è prevista dall'articolo 28, che introduce il nuovo articolo 270-*bis* del codice di procedura penale, attraverso il quale si dispone che, quando l'autorità giudiziaria abbia acquisito, tramite le intercettazioni, notizie riguardanti comunicazioni tra operatori dei Servizi medesimi, deve immediatamente trasmettere al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi nel corso del processo e chiedere se alcune di queste siano coperte dal segreto di Stato. Ritengo che l'introduzione di questa norma sia stata correttamente prevista, in quanto spesso, in questa società ove continuamente ormai siamo osservati e spiati, veniamo a conoscenza di episodi, fatti e notizie unicamente tramite le intercettazioni telefoniche, creando dei veri e propri scandali nazionali, con sentenze di condanna espresse dall'opinione pubblica senza attendere la sentenza degli organi giudiziari preposti in danno delle persone intercettate. Proprio perché episodi come questi potrebbero compromettere la sicurezza dei cittadini, condividiamo la volontà di prevedere una maggior tutela e garanzia non solo per i soggetti coinvolti nelle intercettazioni, ma soprattutto per la tutela del sistema Paese. Altra novità della riforma è la nuova disciplina del segreto di Stato che limita l'utilizzo di questo istituto ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per la tutela della sicurezza della Nazione. Il Presidente del Consiglio ha la possibilità, infatti, di disporre la cessazione anticipata del vincolo, quando sono venute meno le esigenze che ne hanno determinato l'apposizione. Ulteriore importanza è data dalla introduzione del limite temporale al vincolo di segretezza, che cessa quando sono decorsi quindici anni dalla sua apposizione, ma, con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio, si può disporre la proroga del vincolo anche più di una volta. L'articolo 39 del disegno di legge indica anche il limite massimo di durata del segreto, che non potrà non potrà superare i trent'anni, previsione che oggi non sussiste. Novità di grande rilievo è la previsione secondo la quale in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale, affidando alla Corte stessa, nell'ambito del giudizio per conflitto di attribuzione, il compito di contemperare i diversi interessi, pubblici o privati, che possono concretamente entrare in conflitto con le esigenze di tutela del segreto di Stato. Vi è, inoltre, la previsione di un parallelo rafforzamento della funzione di controllo parlamentare grazie al quale è possibile contenere il rischio di abusi o deviazioni dell'operato dei Servizi. In particolar modo, si attribuiscono al Comitato parlamentare, cosiddetto COPACO, poteri e competenze più ampi di quelli attualmente previsti che permetteranno un controllo sull'attività di *intelligence* in tutti i suoi aspetti, compresi quelli operativi, gestionali e contabili. Ciò si è reso più che mai opportuno anche alla luce di recenti episodi verificatisi nel nostro Paese. Desidero ricordare ancora che il nostro Paese, al fine di fronteggiare maggiormente le diverse situazioni di pericolo che possono derivare sia dall'ambito nazionale che internazionale, opera sempre più in un contesto di alleanza, sia atlantica che europea, ma comunque sempre nel quadro di operazioni multinazionali sotto l'egida dell'ONU. Proprio per questi motivi occorre che la nostra struttura di *intelligence* sia al passo con i tempi, con gli strumenti e le strutture dei nostri alleati, al fine di costituire una struttura informativa omogenea e compatta. Bene ha fatto la Commissione a chiarire meglio l'espressione «carattere tecnico militare e di polizia militare» riferita ai compiti esclusivamente svolti dal RIS, così come era stato richiesto dal capo di stato maggiore della difesa ammiraglio Di Paola, aggiungendo «e in particolare ogni attività informativa utile al fine della tutela dei presìdi e delle attività delle Forze armate all'estero» specificando meglio così i compiti, le funzioni ed i limiti di azione. In conseguenza di queste riflessioni, ritengo che il disegno di legge al nostro esame rispecchi e soddisfi, nel miglior modo possibile anche se in maniera non totalitaria, le diverse esigenze che sono state dibattute e rappresentate, creando una sorta di equilibrio che ulteriori modifiche del testo in esame porterebbero a rendere vano ogni sforzo compiuto finora. Ritengo in ogni caso che queste norme avranno l'efficacia auspicata se, come nel passato, pur nel contesto di scenari sempre mutevoli, ci troveremo di fronte a degli operatori che nel loro agire sapranno mettere al primo posto l'interesse dei cittadini e della Nazione.

il disegno di legge in discussione incide su una materia particolarmente rilevante ai fini della configurazione realmente democratica del nostro ordinamento, quale Stato di diritto retto dal principio di legalità. Il tema dei Servizi per l'informazione e la sicurezza implica, infatti, la necessità per il legislatore di stabilire il bilanciamento più equo e garantista possibile tra contrapposte esigenze, quali sono l'azione dei Servizi, tesa a prevenire la commissione di reati suscettibili di minare la sicurezza, e l'assetto costituzionale dell'ordinamento, da un lato, e la natura effettivamente democratica delle istituzioni, dall'altro. È bene, quindi, sottolineare la sinergia imprescindibile tra sicurezza e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali che non possono mai essere sacrificati in nome della prima. Leggere, infatti, quei diritti che per secoli hanno garantito tutti dalla violenza del potere come inutili formalità conduce all'autoritarismo e alla negazione dei principi del costituzionalismo moderno nati dall'esigenza di coniugare giustizia e legalità, eguaglianza e dignità, umanità e politica. Il disegno di legge in esame si muove tra l'esigenza di sicurezza, da un lato, e la tutela dei diritti e dei principi fondativi dello Stato di diritto, dall'altro. Nel complesso, il bilanciamento realizzato risulta in linea di massima condivisibile e pertanto il nostro Gruppo voterà a favore. Resta, tuttavia, da sottolineare come si sia tentato un'ulteriore miglioramento in senso maggiormente garantista del disegno di legge rispetto al suo testo originario, in particolare, attraverso l'esame del provvedimento in Commissione, sia in sede referente che in sede consultiva. Sotto il primo profilo un deciso miglioramento del testo è derivato dall'accoglimento di alcune proposte emendative, anche del nostro Gruppo, volte a valorizzare e garantire con maggiore forza il principio della leale collaborazione tra autorità giudiziaria e Servizi, dal momento che gli organi di sicurezza spesso si trovano ad operare per la prevenzione di reati sui quali contestualmente indaga la magistratura inquirente. Per evitare sovrapposizioni, o casi di violazione delle reciproche attribuzioni, gli emendamenti accolti in Commissione hanno precisato che la collaborazione tra autorità giudiziaria e Servizi non può mai risolversi in una prevaricazione di questi sulla prima, anche al fine di garantire il rispetto del segreto istruttorio e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura sancito dall'articolo 101 della Costituzione. Si tratta di una precisazione importante, soprattutto alla luce delle carenze che la disciplina attuale, di cui alla legge n. 801 del 1977, ha dimostrato nella prassi. Infatti, la normativa prefigura un sistema destinato in teoria a svolgere i propri compiti informativi e di sicurezza nel sostanziale rispetto della legalità e nell'assoluta preclusione di ogni possibile interferenza con il sistema giudiziario. Tuttavia, la prassi ha dimostrato le lacune e le contraddizioni di questa disciplina, che è stata spesso violata, soprattutto nella parte in cui impone ai direttori del SISMI e del SISDE di trasmettere agli organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati e dalle indagini giudiziarie sono emerse gravi torsioni delle norme operative e del modello organizzativo e funzionale dell'attività dei Servizi segreti che accreditano la vulgata sulle deviazioni degli apparati di sicurezza, ma soprattutto la recente vicenda del sequestro di Abu Omar, dei cosiddetti voli segreti, ha dimostrato ancora una volta i limiti e le contraddizioni della disciplina del segreto di Stato, oltre che della sua concreta applicazione, rivelando in senso più generale tutta la fragilità del sistema normativo vigente in materia di organizzazione e funzionamento dei Servizi segreti, svincolati a tal punto da un effettivo e rigoroso controllo politico, da poter impunemente violare anche quelle scarne norme di disciplina dettate dalla legge n. 801 del 1977. È chiaro, quindi, che il maggiore rigore cui si ispira la disciplina del disegno di legge in discussione rappresenta un'importante novità sul terreno delle garanzie e del rispetto delle reciproche sfere di attribuzione degli organi statali. In questa prospettiva garantista, si muove anche il parere reso in Commissione giustizia in sede consultiva che precisa alcuni requisiti e parametri fondativi cui orientare il bilanciamento tra esigenze di sicurezza ed efficacia dell'azione preventiva dei Servizi da un lato, e dall'altro rispetto dei principi di legalità, garanzia del diritto alla difesa e subordinazione dell'operato dei Servizi al controllo parlamentare. In questa prospettiva si muovono anche alcuni emendamenti proposti dal nostro Gruppo nella direzione di un ampliamento dei poteri di controllo e di indagine del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (questa la nuova denominazione del COPACO), cui sono stati attribuiti alcuni dei poteri previsti dall'articolo 82 della Costituzione, limitatamente alle audizioni a testimonianza, al fine di renderne più efficace il sindacato ispettivo, nel quale si esprime il principio di responsabilità politica dell'azione dell'Esecutivo di fronte all'organo rappresentativo della sovranità popolare. Nella stessa prospettiva, si è inteso sancire il divieto di stipula di trattati internazionali in forma segreta, al fine di garantire il coinvolgimento e il controllo dell'organo parlamentare nell'attività di politica estera, senza eccezione alcuna. Sotto un diverso profilo, si sono proposti emendamenti volti ad esempio a restringere l'area di impunità per gli agenti dei Servizi escludendo la scriminante della garanzia funzionale per reati particolarmente gravi, non potendosi ammettere, se non in misura limitatissima ed eccezionale, che lo Stato legittimi la commissione da parte dei suoi funzionari di delitti che altrove sanziona, peraltro con pene pesanti. Altri emendamenti mirano poi a garantire maggiormente il diritto alla difesa dell'imputato o indagato che necessiti di produrre atti o dichiarazioni coperte da segreto, al fine di dimostrare la propria innocenza; tale emendamento traduceva un assunto incontrastato nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il diritto alla difesa e la presunzione dell'innocenza, in quanto appartenenti a quei principi supremi dell'ordinamento, sottratti persino alla revisione costituzionale, non sono suscettibili di limitazione alcuna, neppure in nome della tutela del segreto di Stato. Proprio in quanto legata all'azione di sicurezza dal nemico, l'attività dei Servizi segreti rischia di rifarsi nella sua logica alla prevalenza della ragion di Stato sulle regole dello Stato di diritto, come quando si sancisce l'impunità per gli agenti dei Servizi che commettano delitti anche gravissimi in nome di una non meglio precisata esigenza di difesa dello Stato da possibili nemici, insindacabile perché spesso coperta dal segreto, appunto, di Stato. Vicende recenti ci hanno dimostrato la pericolosità di una simile logica e soprattutto i rischi connessi ad una confusione tra tutela dello Stato e difesa dell'ordine e del potere costituito. È questo il rischio di una lettura dell'azione dei Servizi che noi abbiamo inteso contrastare con forza, intervenendo con proposte migliorative su questo disegno di legge. Perché è importante precisare che la lettera della legge nel definire, oggi come ieri, quale fine dei Servizi "la difesa dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione" intende per "Stato" non certo la compagine di Governo e l'assetto dei poteri costituiti, ma l'ordinamento costituzionale quale sistema di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali. È bene ribadirlo, come abbiamo tentato di fare anche con le nostre proposte emendative.

a nessuno sfugge la constatazione che l'equilibrio tra l'organizzazione dei Servizi di informazione, la disciplina del segreto di Stato e la Carta Costituzionale costituisca la premessa e la condizione perché le relative leggi possano assicurare un sufficiente e rassicurante livello di democrazia nel nostro Paese. Il secondo parametro che deve ispirare che deve ispirare la normativa su sicurezza e segreto di Stato attiene, senza alcun dubbio, alle scelte che Governo e Parlamento devono fare con l'obiettivo di assicurare la pienezza all'esercizio dei diritti dei cittadini accanto all'adempimento dei doveri: ricordava questo stesso concetto il collega Grassi.

sulla stessa linea si pone il disegno di legge in discussione, già approvato dalla Camera dei deputati, che si caratterizza anche per il maggiore rilievo che riserva al sistema di sicurezza, soprattutto sul versante internazionale. D'altra parte, la nuova legge non poteva non tenere conto del nuovo quadro internazionale e della globalizzazione dei fenomeni terroristici, dopo il drammatico attacco alle due torri di New York. Ricordo ancora un magnifico intervento del professor Vittorio Grevi di alcuni anni fa, che inquadrò correttamente il tema della sicurezza del segreto di Stato nella cornice dello Stato di diritto liberale e democratico. Posso dire che il disegno di legge in discussione si colloca anch'esso nella cornice del nostro ordinamento statale di oggi, caratterizzato dalla logica della legalità e dalla forte esigenza di garanzia per le libertà individuali e istituzionali. Le disposizioni dell'articolo 1 del provvedimento, infatti, sottolineano questa necessità laddove assegnano alla Presidenza del Consiglio la direzione e la responsabilità della politica di informazione per la sicurezza nell'interesse della difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste a base della nostra Costituzione. Va anche osservato che con la nuova legge si rafforza il principio delle finalità prevalentemente difensive e non offensive di tutti gli apparati, delle strutture e del personale del sistema dei Servizi di sicurezza. In questa logica viene disciplinata con norma più precisa la regolamentazione del segreto di Stato, accanto alla normativa della sicurezza, entrambe comunque sottoposte ai limiti che derivano dalla scelta che lo Stato ha fatto di interpretare i princìpi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale come punto di equilibrio tra diritti di libertà e democrazia e limiti da essi derivanti e mai superabili o eludibili, neppure con l'esaltazione del sovrano interesse dello Stato. Personalmente, dalla prima lettura del disegno di legge in esame, avevo avuto qualche perplessità sul fatto che la disciplina del sistema di sicurezza dovesse contenere anche la regolamentazione dell'istituto del segreto di Stato che, come è noto, riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e non solo l'apparato di sicurezza. Poi, dall'esame più approfondito e complessivo del provvedimento e soprattutto meglio cogliendo lo spirito che ha animato le scelte della Camera, ho dato l'adesione al disegno di legge anche nella parte relativa alla disciplina del segreto di Stato che non nego presenta ancora oggi una farraginosità che successivamente potrà essere superata. Posso dire che sono stato convinto anche dalle disposizioni all'articolo 17 del disegno di legge, che definiscono in maniera più rassicurante l'ambito di applicazione delle garanzie funzionali, che è il cuore poi di questo disegno di legge, che costituiscono il punto centrale della legittima autorizzazione di eccezionali condotte indispensabili di volta in volta alle finalità istituzionali dei Servizi di *intelligence*. Valgono, tuttavia, i limiti di speciali cause di giustificazione previste analiticamente nei commi degli articoli 17, 18 e 19 del disegno di legge, che definiscono un quadro complessivo di maggiore garanzia per gli operatori di sicurezza, ma anche nello spirito del principio della legalità. Gli obiettivi del disegno di legge di determinare attraverso i Servizi di sicurezza e l'istituto del segreto di Stato un forte sistema di difesa della sicurezza dei cittadini delle istituzioni statali vengono realizzati prevalentemente da un più moderno sistema di *intelligence*, efficiente e determinato nella sua attività, superando le soluzioni di mediazione cui si è ricorso purtroppo nel passato per le differenti posizioni e divisioni delle forze politiche che, sia pure per aspetti limitati, non hanno consentito una più forte funzionalità dei Servizi di sicurezza. Non vanno dimenticate le recenti polemiche sul segreto di Stato, che spesso hanno dato la sensazione che tale istituto non abbia il nobile scopo di aumentare la sicurezza del sistema, ma solo favorire uno schieramento politico e che ciò non è solo sbagliato ma anche profondamente ingiusto. Il disegno di legge, pur accettando il principio della dualità del sistema di informazione per la sicurezza, in qualche modo sceglie la strada di un maggiore accentramento dei poteri dell'organo, costituito dal dipartimento preposto all'armonizzazione e al collegamento dei due Servizi operativi - come ha ricordato poco fa il collega Ramponi - sia pure con concordate scelte correttive nell'esame del disegno di legge in Commissione. Appare rafforzato il ruolo di garanzia del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, che viene disciplinato negli articoli da 30 a 37, con il compito di verificare in maniera continuativa che l'attività del sistema si svolga nel rispetto della Costituzione, delle delle leggi, nell'interesse esclusivo e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Ci siamo molto soffermati nell'esame del provvedimento sulla scelta di assegnare a molti decreti delegati l'attuazione delle norme di principio e di organizzazione e funzionamento dei vari organi del sistema di sicurezza. La scelta è doverosa per la delicatezza degli argomenti, ma mi piace ricordare che in Commissione è stato unanime l'orientamento di assegnare ad un apposito *forum* la vigilanza e il controllo sui processi legislativi che determineranno i decreti delegati, veri cardini della nuova disciplina legislativa del sistema della sicurezza dello Stato. Alcune osservazioni finali. Anche in questo disegno di legge si mantiene costante l'equilibrio tra operare con serenità in segretezza e l'effettivo controllo democratico sull'apparato dei Servizi. Rimane la distinzione che il controllo non può essere cogestione, ma solo conoscenza conoscenza e vigilanza. Il rafforzato ruolo del COPACO mantiene questo limite, senza dar luogo a conflitti di interesse. Il nuovo ordinamento delle garanzie funzionali e degli operatori dei Servizi tiene conto dell'esperienza passata con il vigore della legge n. 801 del 1971, ma dà ragione alle esigenze che la situazione oggi impone, sottolineando la necessità di non lasciare disarmato giuridicamente i nostri operatori della sicurezza di fronte a nemici o avversari più agguerriti e protetti dalla legislazione dei loro Paesi. In questo nuovo quadro un aiuto importante può venire dalla magistratura, che spesso ha avuto nel passato un approccio preventivo nei confronti degli operatori della Sicurezza, dimenticando che si tratta di servitori dello Stato nell'interesse della sicurezza delle persone e delle istituzioni democratiche del Paese. ne parlo io): sono state accolte dal Governo alcune preoccupazioni relative al trattamento economico. L'adesione dei relatori ha consentito una soluzione in questo settore e anche in materia di formazione che pone la normativa allo stesso livello delle altre democrazie del mondo. Onorevoli senatori, onorevoli Sottosegretari, voglio chiudere questo mio intervento testimoniando testimoniando il clima costruttivo registrato nella Commissione referente, anche per l'attenzione costante e intelligente dei rappresentanti del Governo e dei relatori, senatori Pastore e Sinisi. Desidero anche ringraziare i nostri responsabili dei Servizi di sicurezza di ieri e di oggi, tutti gli operatori che anche mettendo in pericolo la loro vita - ricordo il sacrificio di Calipari - hanno lavorato per la sicurezza del nostro Paese, che anche grazie a loro sacrificio non ha subito attacchi ed attentati come è successo in altri Paesi del mondo. Onorevoli senatori, libertà e sicurezza non sono istituti tra loro inconciliabili e incompatibili, se uno Stato liberale e democratico riesce a godere della fiducia dei cittadini. Il Parlamento e il Governo devono impegnarsi in questa direzione. Questa legge che ci accingiamo ad approvare è un esempio di convergenza di analisi e decisione. Speriamo che anche in altri settori si possano registrare intelligenti e necessarie condivisioni che sono indispensabili per il bene del nostro tormentato Paese.

fino al 3 agosto. La seduta pomeridiana di oggi, anticipata alle ore 16, si aprirà con le comunicazioni del Ministro degli affari esteri in materia di politica estera con particolare riferimento allo stato delle missioni internazionali. Nella discussione generale potranno intervenire i Gruppi per 10 minuti ciascuno (15 minuti al Gruppo Misto). Dopo la replica del Ministro avranno luogo le dichiarazioni di voto (10 minuti per ciascun rappresentante dei Gruppi, 15 minuti al Gruppo Misto). Ulteriori proposte di risoluzione e eventuali riformulazioni potranno essere presentate nel corso della discussione generale entro un'ora dalla conclusione delle comunicazioni del Ministro. Tenuto conto della ripartizione dei tempi così definita, le votazioni si concluderanno questa sera, presumibilmente intorno alle ore 21. Domani mattina riprenderà la discussione del disegno di legge di riforma del sistema di informazione e sicurezza. Le due sedute di domani pomeriggio e di giovedì mattina saranno dedicate all'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi per complessive 9 ore. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo potranno essere presentati entro un'ora dall'espressione del parere favorevole da parte del rappresentante del Governo. Non appena trasmesso dalla Camera dei deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia finanziaria - che la Camera prevede di concludere entro la mattinata di domani sarà immediatamente assegnato alla 5a Commissione permanente, che dovrà riferire all'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 31 luglio. Le Commissioni in sede consultiva esprimeranno i propri pareri entro le ore 17 di lunedì 30 luglio. La discussione in Assemblea inizierà nella seduta pomeridiana di martedì 31 luglio. Resta poi inteso che, nella Conferenza dei Capigruppo prevista per martedì 31 alle ore 12, saranno definiti i tempi di esame del decreto-legge in materia finanziaria, gli orari effettivi delle sedute e gli eventuali altri argomenti da inserire nel calendario della prossima settimana che dovrebbe concludersi entro la giornata di giovedì 2 agosto e, se necessario, nella seduta antimeridiana di venerdì 3.

dopo anni di calvario, dopo aver più volte chiesto che gli fosse staccato quel tubo della ventilazione che proseguiva, con evidente accanimento terapeutico, una vita per lui diventata impossibile, come per Welby. Se ne è andato così e ora non importa come, se essendosi negato cibo e acqua negli ultimi giorni o se per consunzione, estenuazione, inedia. Se ne è andato, e davanti a casa sua c'erano i carabinieri. Erano arrivati a metà luglio. A controllare che cosa? Chi? Non certo i movimenti di chi non poteva neppure muoversi, parlare, ma a cui era consentito solo un battere di ciglia. Ma un giudice a cui Nuvoli aveva chiesto di poter morire glieli aveva messi sotto casa quei carabinieri, perché ci sono medici che potevano alleviare le sue sofferenze e questo non lo dovevano fare, quella soglia non la dovevano varcare. I carabinieri stavano lì esattamente a piantonare un morente. L'articolo 32 della Costituzione, che stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento, è stato semplicemente ignorato. Se ne è andato, però, in un giorno non qualunque: poche ore prima, un altro giudice, una donna, aveva deciso che a certe condizioni la richiesta di un malato di rifiutare le cure è un diritto e che la risposta del medico è un dovere. È troppo tardi per lui ormai, ma forse non è troppo tardi per altri. Ci auguriamo che il Parlamento trasversalmente - non è certo una questione di schieramenti - legiferi su questa materia materia e che la politica riacquisti la sua autonomia e la sua forza, prima che per i diritti di ciascuna persona, per la dignità dei morenti.